ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 3 febbraio. febbraio. Per la settimana in corso resta confermato l'esame dei disegni di legge concernenti il condominio degli edifici, l'Ordine della Stella della solidarietà italiana e il personale degli uffici consolari. Lo svolgimento del sindacato ispettivo è stato anticipato alla seduta antimeridiana di giovedì 27 gennaio. Pertanto la seduta pomeridiana di giovedì prossimo non avrà luogo, anche al fine di consentire più ampi spazi di lavoro alle Commissioni impegnate nell'esame del decreto-legge recante proroga di termini legislativi. Le sedute della prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 1° febbraio, saranno prevalentemente dedicate alla discussione del disegno di legge comunitaria 2010, nonché all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi nel corso di questa settimana.

proposte parlamentari, che avevano già avuto un loro sviluppo e approfondimento nella scorsa legislatura. In questa legislatura ci si è avvalsi anche dei lavori che avevano portato a un testo condiviso nella scorsa legislatura, e i lavori della Commissione sono stati quindi impostati nel senso delle conclusioni e degli approfondimenti cui si era già pervenuti. Si cerca di dare delle risposte in termini di attualità ad un problema problema abbastanza antico, materia di approfondite discussioni, e non puntualmente definito dal nostro codice civile, anche in considerazione del fatto che i problemi inerenti alla materia condominiale hanno avuto un'accelerazione ed una implementazione notevolissima nel corso degli anni, determinando un contenzioso enorme; basti pensare che coinvolti dalla materia condominiale sono 40 milioni di cittadini, ossia 12 milioni di famiglie. È una delle ragioni di maggiore aggravio del contenzioso in materia civile. che si propone all'Assemblea si cerca di andare incontro alle esigenze scaturenti da alcune imperfezioni e dall'incompletezza della normativa. Alcuni punti rimangono sicuramente in sospeso, in quanto è stato difficile trovare il giusto equilibrio su alcune posizioni. Dispiace, essendosi in Commissione proceduto a numerose audizioni, che ancora oggi si siano levate delle voci dissonanti, a dire il vero non espresse durante le audizioni.

Se fossero arrivate delle altre sollecitazioni, anche dagli interessati, probabilmente il testo poteva essere, non so come, ma di più alto profilo. Abbiamo cercato di raccogliere i contributi da parte di tutti, ed il provvedimento offerto sicuramente risolve alcuni problemi. Probabilmente, su alcune questioni ci potrebbe essere una lievitazione del contenzioso, ma su molte altre il contenzioso verrà disciplinato in maniera più soddisfacente. Quindi, sull'impianto generale e sull'articolato proposto, sicuramente, come Italia dei Valori, riteniamo soddisfacente il punto di approdo. Valuteremo gli emendamenti proposti e la possibilità di prenderli in considerazione. Comunque il testo proposto è frutto di un lavoro comune, condiviso, fatto con serio approfondimento. E di questo bisogna anche ringraziare il senatore Mugnai che si è fatto carico di coordinare i diversi testi.

Non sarebbe stato sufficiente e opportuno unificare e rendere omogenea la normativa già esistente, dispersa nei rivoli della farraginosa regolamentazione nazionale, al fine di consentire una più fruibile lettura della stessa? Noi crediamo di sì. Invece, ancora una volta, si persevera nella pseudoriforma, peraltro affatto condivisa, solo per fregiarsi dell'approvazione di un nuovo intervento normativo e propagandarlo come rivoluzionario, innovativo. Tutto questo, senza badare alle conseguenze. Fin dall'inizio il dibattito si è concentrato sulla proposta di trasformare il condominio da ente di gestione a soggetto dotato di personalità giuridica. Proposta che poi si è tradotta in un nulla di fatto. Questa riforma non è affatto ambiziosa: oserei definirla di basso profilo. Provocherà, infatti, maggiori costi per i condomini, senza alcun beneficio per gli stessi. Basti considerare la figura dell'amministratore, i cui requisiti assomigliano più a quelli richiesti ad un amministratore delegato che a quelli di un mero mandatario: un'impostazione le cui conseguenze ricadranno ancora una volta sulle tasche della collettività. Il nostro impegno sin dall'esame in Commissione è stato orientato *in primis* a tutelare il cittadino, soprattutto il piccolo proprietario, salvaguardandolo dall'eventuale rincaro dei costi di gestione conseguenti alle modifiche che si vogliono introdurre. In secondo luogo, con le nostre proposte abbiamo puntato sulla necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionalmente riconosciuti e di assicurare l'armonizzazione del testo con la disciplina ordinaria esistente. Ci siamo preoccupati, insomma, di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, alla luce dei troppi, frequenti, drammatici fatti di cronaca, cercando di rafforzare le misure necessarie a vigilare sulla staticità degli edifici. In particolare, mi riferisco alla nostra proposta relativa all'istituzione di un registro del fabbricato nelle zone sismiche, ove annotare le modifiche strutturali succedutesi negli anni sulle singole unità abitative e sul complesso dell'immobile. Ciò avrebbe permesso di avere un «diario» degli interventi, allo scopo di evitare, col tempo, il sovrapporsi nelle strutture di azioni Prendiamo atto che alcune delle nostre iniziative sono state accolte in Commissione. Il forte impegno del nostro Gruppo ha dato i suoi frutti sul fronte della salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, che garantisce la proprietà privata, scongiurandone Non altrettanta sensibilità si è dimostrata nei confronti delle nostre proposte volte a garantire nel condominio la certezza della stabilità dei fabbricati, specie quelli di vecchia costruzione. Nonostante il nostro contributo, dobbiamo ancora registrare una contraddittorietà nell'ambito della stessa proposta ed una scarsa armonizzazione di questa con la normativa corrente. Non abbiamo condiviso, in quanto lesivo della *privacy*, un gravoso meccanismo di pubblicità a carico dell'amministratore, i cui requisiti, previsti dalla normativa che si va ad introdurre, rendono di fatto più difficile rendono di fatto più difficile l'accesso alla professione. Crediamo, al contrario, che, visti gli elevati tassi di disoccupazione soprattutto tra i giovani, si dovrebbe potenziare e promuovere l'accesso al lavoro dei più giovani, e non ostacolarlo. Né abbiamo condiviso che l'annotazione in un registro presso la camera di commercio potesse legittimare l'attività, fino al punto da considerare inadeguata la professionalità di chi invece è iscritto in albi e collegi professionali previo esame di Stato ed è certamente all'altezza di ricoprire questo ruolo. Altrettante perplessità hanno suscitato in noi le complesse incombenze e sanzioni previste, specie sugli adempimenti a carico dell'amministratore, che appaiono eccessive e demotivanti giacché presentano degli ostacoli che complicano non poco l'attività e inducono i professionisti ad accettare l'incarico solo dietro compensi elevati. Ciò determina un incremento dei costi per la proprietà in condominio, già oppressa da recenti aumenti delle spese per servizi e forniture. Come anticipato, alcune nostre proposte emendative al testo, che in Commissione in un primo tempo la maggioranza insisteva così fieramente nel respingere, sono state ragionevolmente accolte, e ciò va riconosciuto, oltre che al nostro impegno nell'interesse della collettività, anche alla sensibilità del relatore, della quale voglio dare assolutamente atto. atto. Le modifiche da noi proposte che sono state accolte non sono state però sufficienti a dissipare del tutto quelle disarmonie che permangono nel testo. Ci auguriamo, quindi, che l'odierno passaggio in Aula, da noi fortemente voluto per consentire una più ampia e condivisa disamina del provvedimento, contribuisca a correggere la proposta, a salvaguardia dell'interesse del cittadino. *(Applausi

come è già stato detto, si conclude oggi, per quanto riguarda il Senato, il tentativo di riformare l'istituto

Voglio ricordare che la disciplina di questo istituto è contenuta nel codice civile, quindi in una normativa che risale al 1942 e che è alla soglia del compimento del 70° anniversario.

Grazie

È vero, è già stato ricordato, che molta parte della discussione che attiene a questa riforma ha riguardato la questione della personalità giuridica: se attribuire o meno

La proposta che noi approveremo in queste ore ha dato una risposta negativa. Non si è ritenuto di trasformare, come dicevo prima, questo istituto, che è una comunione di proprietari, in una

di prevedere una opzione per il condominio verso questa forma giuridica non sfuggendoci, peraltro, che l'istituzione di un sistema duale non renderebbe facile ai terzi capire

di essere ulteriormente esaustive rispetto alle questioni poste. Al di là di questa vicenda, che - come dicevo - ha occupato buona parte della nostra discussione, nostro esame contiene notevoli cambiamenti; non è una riforma qualsiasi. Tali cambiamenti partono da una modifica sostanziale dei *quorum* deliberativi delle assemblee, una delle questioni che nella vita comune

L'intero regime delle trascrizioni viene sostanzialmente modificato a tutela degli interessi sia di chi acquista, che dei terzi in generale.

che il proprietario mostri dei certificati, ma vi è la possibilità per l'amministratore che venga sollecitato attraverso una procedura all'uopo definita di entrare nell'unità abitativa a vedere se davvero sussistono ragioni di pericolo.

una realtà che di certo dal 1942 ad oggi ha conosciuto modifiche e novità di un certo tenore e di una certa importanza.

e trovare anche forme e modi di adeguamento di strutture e di unità abitative alle esigenze della vita di tutti. *(Applausi

in particolare i colleghi del Comitato ristretto, che hanno dimostrato grande interesse per l'argomento in discussione quest'oggi e che con grande competenza hanno sviluppato un disegno di legge coerente rispetto a quella che è stata la nostra proposta iniziale. Come sappiamo, le norme in materia di tenuta del registro in cui viene annoverato il nominativo dell'amministratore del condominio, cosi come viene menzionato negli attuali articoli 1129 e 1138 del delle disposizioni di attuazione del codice civile, non hanno mai trovato una effettiva applicazione. Pertanto, con il disegno di legge da me proposto prevedevo l'istituzione effettiva di tale registro da tenersi presso l'Agenzia del territorio. Ritengo opportuno, quindi, fornire un dato a supporto dell'importanza di questa modifica. La direzione studi e ricerche economico-fiscali del Ministero dell'economia ha identificato, a tutto il 2009, in base al trattamento dei codici fiscali intestati ad ogni condominio, ben 1.018.821 condomini e 334.317 amministratori. L'esigenza di un registro in cui vengano annoverati i nominativi di coloro che svolgono la professione di amministratore di condominio, peraltro già previsto dal codice civile, è quindi forte, se consideriamo il notevole incremento del numero degli edifici condominiali, nonché il fatto che non esiste un'unica associazione professionale dei proprietari di fabbricati. Come già proposto nella XV legislatura dal senatore Pastore e da altri colleghi, attraverso il disegno di legge Atto Senato n. 6, dal Comitato ristretto della Commissione giustizia il 27 novembre 2006, e come indicato nel disegno di legge che mi vede primo firmatario, il registro potrebbe essere tenuto dall'Agenzia del territorio, dall'Agenzia del territorio, la quale si è dichiarata disponibile a garantire una gestione più omogenea del registro degli amministratori su tutto il territorio nazionale, colmando così un vuoto normativo inspiegabilmente ignorato da molto tempo.

i cui costi dovranno essere sostenuti dagli amministratori di condominio, quelli che ne richiedono l'iscrizione, come avviene in Francia, per esempio, presso il registro prefettizio, o nei registri tenuti presso le camere di commercio in altri Paesi europei. Il registro andrà ad affiancarsi ai tradizionali registri immobiliari al momento gestiti dagli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. In questo modo verrà garantita, attraverso sistemi informatici, la conoscibilità dei rappresentanti legali e delle amministrazioni condominiali. Tutto ciò favorirebbe il perseguimento di interessi pubblici rilevanti sia nell'ambito fiscale, sia in quello della sicurezza, in quello del risparmio energetico, dell'ambiente, nonché della protezione civile. L'Agenzia del territorio potrà avere a disposizione un utile riferimento di collaborazione ai fini della realizzazione dell'anagrafe immobiliare integrata sia per i beni comuni censibili, sia per il contrasto ai fenomeni di evasione-elusione fiscale. Mi auguro una rapida approvazione

Sarà dunque una grande prova per tutti. La speranza è quella di avviare un sistema unitario che garantisca una più efficiente gestione di un settore che da tempo attende miglioramenti. *(Applausi dal Dichiaro chiusa la discussione generale.

è stato, e tuttora continua ad essere, nelle sue implicazioni giuridiche, una delle fonti principali di contenzioso per quanto riguarda la materia civile, e che quindi necessariamente deve essere affrontato

è sottoposto all'Aula e che certamente - condivido il ragionamento del collega Galperti - non sarà la migliore in assoluto delle riforme, ma di sicuro rappresenta la migliore delle riforme possibili,

Una questione, forse più delle altre - al riguardo credo sia giusto soffermarsi un istante - ha lungamente impegnato, prima i componenti del Comitato ristretto,

attribuire al condominio distinta personalità (perché di ciò poi in realtà si tratterebbe: non della capacità giuridica, posto che il condominio già oggi ha la capacità giuridica, in quanto l'amministratore lo rappresenta), che trova ancora un'eco, sia pure in una forma diversa rispetto a quella inizialmente prospettata, in uno degli emendamenti del collega Legnini, cui ha fatto riferimento anche il senatore Galperti. Da questo punto di vista, voglio rimarcare ancora una volta come il tema sia stato affrontato da tutti i componenti del Comitato ristretto anche della Commissione giustizia, senza alcuna pregiudiziale ideologica o giuridica al riguardo, ma semplicemente cercando di valutare se siffatta prospettazione potesse in qualche modo essere organicamente inseribile nel testo che stavamo licenziando e al tempo stesso praticabile senza creare ulteriori distorsioni di sistema.

dove si parla della possibilità di concedere la capacità e, *rectius*, la personalità al condominio per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni. Ciò significherebbe che il condominio diventerebbe soggetto terzo che dispone dell'amministrazione e della conservazione delle parti comuni e, quindi, diventerebbe soggetto titolare di diritti e doveri, obblighi o diritti, in relazione a dette parti. assumerebbe personalità, perché dovrebbe essere munito di un patrimonio: altrimenti, come potrebbe rispondere delle obbligazioni nei confronti dei terzi per quegli atti di amministrazione o conservazione?

condominio di autonomo patrimonio con il quale rispondere si dovrebbe in qualche modo privare i condomini del proprio diritto di comproprietà sulle parti comuni: è evidente che ciò cozza insanabilmente con il principio costituzionale della tutela della proprietà. Per tale ragione, prima

non avesse avuto beni suscettibili di essere separati dalla loro funzione di supporto delle parti comuni (ad esempio, un parco dotato di strutture) e quindi fosse stato suscettibile di autonoma valutazione economica.

chiarezza e decisione, prevedendo una serie di meccanismi per i quali sia possibile accedere all'interno delle singole proprietà e verificare le condizioni nelle quali si trovano quegli impianti

Vi è stata un'accelerazione delle dinamiche della vita condominiale attraverso un passaggio significativo contenuto nell'articolo 1117*-ter*, dove per la prima volta, ma in modo coerente, non solo con l'impianto della legge ma anche con l'impianto normativo in generale, ed in particolare con lo stesso dettato costituzionale, si affronta il problema della staticità della vita condominiale legata al criterio dell'unanimità per quanto riguarda la disposizione delle parti comuni.

sul diritto di proprietà, sia pur nella forma della comproprietà per i condomini, ma meglio si persegue l'utilità condominiale. Credo che questo rappresenti un grande passo in avanti.

per le obbligazioni rispondono prima i condomini morosi, e solo successivamente quelli virtuosi. Si tratta di un'attenuazione, ma è ad ogni modo un significativo passo in avanti verso quella che può essere una tutela assoluta di chi è sempre e costantemente in regola all'interno del proprio condominio. Abbiamo previsto per la prima volta una maggiore responsabilizzazione della figura dell'amministratore, gravandolo anche dell'obbligo di garantire assicurativamente le responsabilità conseguenti alla propria attività. Avevamo pensato qualcosa di più, ma abbiamo anche tenuto oggettivamente conto di uno degli aspetti che il collega Serra ha voluto prima ricordare per quanto riguarda l'avvio alla professione. Certo, la polizza assicurativa non copre la figura dell'amministratore che opera una malversazione dolosa a carico del condominio, questo sia chiaro: sarebbe stata necessaria una cauzione, cosa che sarebbe impossibile prestare, soprattutto per la maggior parte di coloro che accedono oggi alla professione, per evidenti ragioni di garanzie bancarie. Tuttavia, già la polizza assicurativa obbligatoria rappresenta un significativo passo in avanti. Inoltre, l'obbligatorietà del conto condominiale eviterà che vi possano essere confusioni fra le somme di pertinenza del condominio e quelle di pertinenza dell'amministratore, con verifiche da parte dei condomini. Tutto ciò significa oggettivamente

regolamentato la figura del supercondominio e del condominio orizzontale, assolutamente sconosciute, per evidenti ragioni, al legislatore del 1942, ma che oggi sono invece piuttosto diffusi: basti pensare alle villette a schiera, servite da tutta una serie di porzioni comuni che non sono quelle tradizionali del condominio inteso come edificio

che non era possibile, per ragioni legate anche alla normativa europea in materia di professioni non regolamentate, istituire un albo. Tutti si augurano che l'amministratore professionale sia il più professionale possibile: abbiamo istituito un meccanismo che non ha costi per l'amministrazione dello Stato perché è a carico degli stessi amministratori. Si tratta di un registro presso le Camere di commercio, che consente, intanto, un primo positivo effetto di assoluta, immediata evidenza: non solo la tracciabilità degli amministratori professionali, non solo la verifica dell'esistenza o meno di carichi pendenti o di condanne per reati reati contro il patrimonio, che potrebbero in quel modo costituire condizione ostativa, ma anche e soprattutto un virtuoso effetto antielusivo. È infatti evidente che chi si iscrive non potrà certamente operare se non in modo trasparente ed ufficiale. Mi pare che, sia pure nella rapidissima sintesi di alcuni degli aspetti più peculiari, si possa parlare - come altri colleghi hanno ricordato di una riforma alla quale tutti, maggioranza e opposizione, hanno significativamente contribuito e che se non risolverà del tutto la complessa materia condominiale, quanto

una proposta legislativa di riforma del condominio che è il risultato dell'esame meditato e competente svolto dalla Commissione giustizia del Senato. Il testo raccoglie - come è noto - il contributo di diverse iniziative di origine parlamentare, per molti aspetti convergenti verso un unico obiettivo, quello dell'aggiornamento della disciplina civilistica alle nuove condizioni economico- sociali, come ha sottolineato anche il relatore Mugnai. L'unità e la validità dell'impianto che - sulla base di quelle proposte - oggi questa Assemblea è messa in grado di valutare, sono dovute allo spirito costruttivo e non pregiudiziale, che è stato esemplarmente espresso dalla Commissione giustizia nel suo complesso, grazie alla guida sicura del suo Presidente, alla dedizione del suo relatore, senatore Mugnai, e al lavoro di tutti i componenti. Per tutto questo esprimo il convinto e sincero ringraziamento del Governo, che non ha mai mancato di apportare il proprio contributo e la propria adesione nel corso dell'esame. Il testo unitario, approvato dal Comitato ristretto nel febbraio del 2010, è stato discusso in Commissione nel luglio successivo e sottoposto a numerosi emendamenti. Come sempre il testo potrà essere migliorato, ma il punto di sintesi individuato già costituisce, già costituisce, a giudizio del Governo, un importante passo avanti rispetto al regime vigente. Punto di partenza comune di tutte le proposte esaminate è stata infatti l'indifferibile esigenza di adeguare la disciplina civilistica

sono già evidenziate dalla sapiente ed esauriente relazione, che mette in luce le oltre venti modifiche ad articoli del codice civile e di successive disposizioni attuative che la proposta reca. Ne risulta una disciplina più completa e analitica delle parti comuni e del cosiddetto supercondominio, la più efficace tutela delle destinazioni d'uso delle parti comuni e delle proprietà esclusive, un nuovo e più elastico regime delle delibere assembleari concernenti le innovazioni, la puntuale previsione dei il rafforzamento dei poteri dell'amministratore per quanto riguarda l'intervento urgente in caso di rischi per la sicurezza dell'edificio, l'istituzione del registro dell'anagrafe condominiale nonché - presso le Camere di commercio - del registro degli amministratori di condominio. Si tratta di soluzioni in gran parte dibattute nel corso della precedente legislatura, senza che fu possibile però in quella sede giungere all'esito finale. Su esse, pertanto, non mi soffermo oltre. Vorrei solo sottolineare due questioni. In primo luogo, l'importanza non solo di quello che il disegno di legge contiene, ma anche di

la scelta di non approdare ad innovazioni più marcate - con questo rispondo al senatore Serra - non è il frutto di una sottovalutazione di nuovi e possibili orizzonti ma, al contrario, l'esito di una attenta ponderazione di profili più radicali, dalla definizione di una personalità giuridica condominiale all'istituzione di un vero albo professionale. Anche in questo il disegno di legge dà prova di gradualità ed equilibrio. In secondo luogo, evidenzio il valore - indiretto quanto si vuole, ma non per ciò stesso meno decisivo che questa riforma potrà esprimere in termini di riduzione del contenzioso civile, considerata la nota incidenza delle cause condominiali sul complesso della litigiosità tra parti private, e valutato il contributo di chiarezza che questo testo apporta nel settore, valorizzando in termini costruttivi quanto è emerso in questi anni dalla giurisprudenza. La rimozione della cause che ostacolano la fruizione di una giustizia civile degna di questo nome è, oltre che un obiettivo costante di questo Governo, un'esigenza ineludibile di questo Paese. Il conseguimento di questo obiettivo passa per un'azione complessiva e partecipata e, dunque, anche per questo disegno di legge, del quale si raccomanda una convinta ed ampia approvazione.

«La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 5.0.100 parere non ostativo, segnalando al comma 1 che la facoltà di procedere alle innovazioni in materia di barriere architettoniche, anche in deroga ai regolamenti comunali e alle disposizioni urbanistiche edilizie e di decoro architettonico, è suscettibile di ledere l'autonomia riconosciuta agli enti locali; sull'emendamento 30.0.100 parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i commi 6 e 7, in quanto contengono disposizioni di carattere impositivo, lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali; sui restanti emendamenti parere non ostativo».

parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 26, comma 1, quinto capoverso, dopo le parole "forma societaria" siano inserite le seguenti parole:

sulla base di procedure indicate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza biennale al fine di garantire l'equilibrio finanziario relativo alla tenuta del registro. La tenuta del registro non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica". Infine, conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da "e stabilisce" fino alla fine del periodo. In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 26.100, 30.0.100 e 31.0.100, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

inviterei sin da adesso i presentatori degli emendamenti, con alcune esclusioni che mi permetterei di rappresentare, al ritiro degli stessi. Questo, perché essi rappresentano in alcuni casi una mera superfetazione del testo.

il legale rappresentante di un'entità giuridica che può essere centro di imputazione giuridica di rapporti: è qualcosa di meno, una forma attenuata di collettivizzazione degli interessi dei condomini medesimi. Ciò che nel mio emendamento si chiede non è - attenzione il riconoscimento della personalità giuridica che costituirebbe, esso sì, una trasformazione della natura dei condomini troppo spinta, una sorta di trasformazione in organismi societari in cui il patrimonio del condominio sarebbe del tutto autonomo dalla proprietà dei condomini, con quel che segue. Ciò che si chiede è appunto il riconoscimento della capacità giuridica, cioè della possibilità di rendere il condominio autonomo titolare di rapporti giuridici nei confronti dei condomini e dei terzi.

dalla preoccupazione della difficoltà di gestione di un istituto giuridico di questo tipo? Insisto per tenere conto della trasformazione

il senatore Mugnai non sono solo cittadini persone fisiche, ma sono società, titolari di attività economiche e professionali: insomma, tutta la realtà, che conosciamo tutti molto bene, della vita in condominio nel nostro Paese, fonte di impegni e preoccupazioni quotidiani, non solo sotto il profilo finanziario ma anche relazionale, fonte di contenziosi, e tutto ciò che conosciamo.

che possono essere suscettibili di un utilizzo economico autonomo, per esempio gli impianti sportivi. Possono essere titolari di rapporti giuridici complessi: Possono essere titolari di rapporti giuridici complessi: pensiamo ad esempio a tutta la problematica riguardante l'installazione di pannelli solari, impianti di produzione di energia, oggetto di un emendamento successivo a firma dei senatori Della Seta e Ferrante, su cui ritorneremo, cioè la possibilità, per esempio, di poter utilizzare una parte del patrimonio o di poter gestire una parte dei beni comuni in modo autonomo rispetto ai rapporti condominiali in senso stretto e quindi per questa via fare meglio gli interessi dei condomini. È difficile che un grande condominio possa trovare l'intesa, l'accordo, il luogo di decisione, le maggioranze per poter fare operazioni che un condominio munito di capacità giuridica ed un amministratore legale rappresentante, titolare di poteri, di obblighi e di prerogative, può altrimenti fare. Ecco perché questa innovazione, la capacità giuridica del condominio, costituirebbe un elemento di modernizzazione. Peraltro, aggiungo che, per quel che è di mia conoscenza, gran parte degli ordinamenti giuridici europei contemplano queste ipotesi. Quindi, il nostro rimarrebbe uno dei pochi ordinamenti sotto questo aspetto non adeguati ai tempi la personalità giuridica, non è questa forma attenuata, blanda, di imputazione degli interessi e dei rapporti giuridici che conosciamo oggi e che è fonte di molte problematiche per esempio tra l'amministratore e i condomini: è una forma intermedia, in cui in qualche modo si afferma un'autonomia del soggetto giuridico condominio rispetto ai condomini.

Non prevediamo una tipizzazione precostituita di condomini muniti di capacità giuridica: diciamo che se i condomini lo ritengono, secondo le maggioranze previste dalla legge - e dall'emendamento stesso - possono accedere a questa organizzazione giuridica dei loro interessi e dei loro beni. Perché se fosse una disposizione generalizzata, se fosse un obbligo il riconoscere al condominio la capacità giuridica, l'intero impianto della legge dovrebbe essere rivisitato e i condomini sarebbero, sotto il profilo giuridico, qualcosa di diverso da ciò che invece è disciplinato da questo testo normativo. Invece, attribuendo questa facoltà, attribuiremmo a molti cittadini italiani - ma anche a molti titolari di imprese, di attività economiche e professionali - la possibilità di munirsi di uno strumento aggiuntivo che consentirebbe di separare di più la vita quotidiana, spicciola, del condominio rispetto alla gestione, all'amministrazione dei beni del condominio, a volte suscettibili anche di un utilizzo di carattere economico nell'interesse dei condomini medesimi. Questa è la ragione per la quale mi permetto di insistere e chiedo un voto. Naturalmente non è un fatto che cambia radicalmente le cose; sarebbe però un passo positivo nella direzione che mi sono sforzato di spiegare.

il relatore si è ulteriormente convinto della bontà del percorso che prima il Comitato rispetto e poi la Commissione hanno adottato. Cercherò quindi, nel modo più pragmatico e semplice possibile, di spiegare all'Aula perché del genere a maggioranza, ancorché sia ipotizzata come facoltà e non come obbligo. Se noi ipotizziamo un sistema in forza del quale creiamo un soggetto terzo - il condominio che ha la possibilità di istituire autonomi rapporti giuridici con soggetti terzi rispetto al condominio, va da sé che in relazione a questi autonomi rapporti giuridici esso debba rispondere: mi pare un fatto assolutamente evidente. evidente. Ebbene, per poter rispondere, nel momento stesso in cui va a instaurare, per l'amministrazione e la conservazione di parti comuni dell'edificio, rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica - perché di ciò si tratterebbe in larghissima parte - deve essere in grado di farlo. Ne consegue quindi che deve avere un patrimonio (non faccio adesso la disquisizione tra capacità e personalità relativamente al patrimonio). è possibile che, a maggioranza, l'assemblea condominiale costituisca un patrimonio, che evidentemente deve discendere da una sorta di spoliazione del diritto di comproprietà dei condomini dissenzienti rispetto a quella delibera? Questo è il punto. Potrei convenire laddove eventualmente si parlasse di decisione all'unanimità, perché all'unanimità il condominio potrebbe anche, teoricamente, attribuirsi capacità giuridica. giuridica. Si tratterebbe comunque di un'innovazione di non trascurabile entità, perché di fatto daremmo al condominio, soggetto terzo, personalità giuridica. Questa è l'unica ragione per cui comunque rimangono fortissime le perplessità. Nulla esclude che un domani si possa andare verso una direzione che è comunque di una sorta di totale spersonalizzazione di ciò che oggi noi però innegabile il fatto che a maggioranza non sia possibile incidere su un diritto assoluto di proprietà, sia pure nella forma della comproprietà delle parti comuni: questa è l'obiezione

Grazie

la contestazione di un'affermazione del senatore Mugnai, che non condivido nel modo più assoluto. L'attribuzione della capacità giuridica al condominio non significa affatto mettere a rischio le quote comuni dei condomini: neanche per sogno.

nei modi e nelle forme che ho precisato nella mia illustrazione. Quindi, ove fosse questo il timore, sarebbe assolutamente infondato, e comunque non è nostra intenzione

per una ragione ovvia: prevedere infatti che un condominio possa avere una configurazione diversa da un altro perché ciò è voluto dall'assemblea dei condomini mi sembra una soluzione al problema piuttosto piuttosto originale, che non condivido. Se vogliamo parlare di capacità giuridica, anche se non utilizziamo questo termine nella legge, intendiamo comunque un centro di imputazione di diritti, di rapporti giuridici, di obblighi con una sua caratteristica che non deve necessariamente tradursi in una soggettività di diritto ma che in ogni caso ha una sua particolare qualificazione ed una particolare rappresentanza. Essendo convinto che nei condomini, anche dopo questa riforma, sia sotteso il tema della capacità giuridica, ritengo l'emendamento

Anche per noi non era accettabile il contrasto con tutte le altre norme rispetto al parere dell'ufficio tecnico, però abbiamo ritenuto di poter

viene proposto all'emendamento 6.260. Soltanto questa è la ragione dell'invito al ritiro; non ve ne sono altre. È chiaro che un testo che ha l'ampiezza di quello che stiamo trattando entro certi limiti una serie di adempimenti non può che trattarli per capi generali e non in modo assolutamente partitico come questo. Questa era l'unica ragione per l'invito al ritiro.

Grazie

del regolamento di condominio a prescindere dai singoli diritti che lo costituiscono, che sono spesso di natura e configurazione diverse, dando luogo anche a fenomeni di incertezza e di litigiosità che una previsione espressa di trascrizione potrebbe eliminare, come nella prassi e nella pratica corrente si sta operando. La seconda questione riguarda la previsione del regolamento predisposto dal proprietario originario, il cosiddetto regolamento contrattuale, che ormai ha piena cittadinanza nel nostro ordinamento e credo sia anche legittimato dalla riforma.

della pubblicità dei diritti e della litigiosità in materia condominiale, per quanto concerne il tema del condominio.

10.6, devo dire che introduce un criterio eccessivamente rigoroso dal punto di vista delle annotazioni, che potrebbe determinare qualche difficoltà

Grazie

rispetto alla possibilità che anche da parte dei condominii si contribuisca a quei programmi che eventualmente le amministrazioni locali promuovono per il miglioramento delle condizioni di vivibilità del contesto urbano in cui è collocato anche il singolo edificio o condominio. Vorrei però raccomandare al relatore e al rappresentante del Governo, se possibile, una riconsiderazione ed analoga attenzione sull'emendamento 13.101 con il quale si intende intende affrontare un problema di cui ci si occupa troppo poco. Parliamo tutti della sicurezza delle città, dei problemi dell'insicurezza dei cittadini, e su questo si discute, si avanzano proposte. C'è un fenomeno però che non stiamo monitorando adeguatamente: talune problematiche di disagio e di insicurezza dei cittadini, specialmente delle persone più deboli, soprattutto degli anziani, si stanno spostando dai luoghi pubblici delle nostre città alla dimensione degli ambienti di relazione privata, come possono essere i condomini, i luoghi dove si concentrano più famiglie. Ci sono state in questi anni nelle nostre città, in tante periferie, delle trasformazioni; persone persone e famiglie che sono invecchiate nel tempo e che convivono all'interno di un palazzo con nuovi inquilini, che sono magari giovani, che hanno caratteristiche e stili di vita diversi, portatori di esperienze culturali diverse. Questo talvolta genera delle situazioni di estraneità, incomprensione e disagio, che so bene dovrebbero essere risolte dal regolamento di condominio o dalla responsabilità del proprietario, nel caso degli inquilini,

facendo salva ovviamente la competenza dell'assemblea condominiale e il mandato dato all'amministratore di condominio, si propone di introdurre un riferimento in da aprire un terreno di valutazione, di riflessione e di intervento, non perché l'amministratore di condominio debba risolvere tutti i problemi, ma perché possa dare un contributo a disinnescare percorsi che possono determinare tensioni e contraddizioni all'interno della dimensione dimensione delle relazioni condominiali, da cui rischiano di scatenare un senso di frustrazione e di impotenza che incidono significativamente proprio su quella percezione di benessere e di sicurezza a volte, basterebbe pochissimo per cercare di operare positivamente. L'invito quindi è ad una riconsiderazione di una proposta che, secondo me, sarebbe qualificante sotto il profilo proprio dell'arricchimento del profilo, della dimensione,

è - ma nell'ambito di un testo come questo, esso si tradurrebbe sostanzialmente più in una dichiarazione di intenti, sprovvista di una specifica forma di attuazione che si in una sanzione specifica o nella richiesta di un eventuale provvedimento giudiziario a sostegno di quelle eventuali iniziative. *Mutatis mutandis*, è come una di quelle formule che spesso si trovano nella contrattualistica anglosassone

**Il Senato non approva**.

a mio modo di vedere l'introduzione nel nostro ordinamento della possibilità per l'usufruttuario e il conduttore di esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione, alla gestione quotidiana del condominio,

reintroduce, l'approvazione all'unanimità delle tabelle millesimali, laddove la

un profluvio di ricorsi. Noi riteniamo che la maggioranza qualificata sia di per sé sufficiente ad introdurre introdurre un elemento di novità assolutamente in tendenza con il resto della normativa che questo disegno di legge introduce, vale a dire la riduzione delle delle maggioranze, eliminando l'unanimità, che di fatto congela e impedisce un corretto evolversi dei rapporti condominiali. Mi pare strano

argomentando l'impianto, il contenuto e i profili qualitativi del disegno di legge al nostro esame, ha spesso sottolineato il fatto che con questa disposizione normativa si introduce un miglioramento dal punto di vista delle regole, delle procedure procedure da seguire anche sotto il profilo dell'esercizio dell'attività professionale dell'amministratore di condominio. L'emendamento da me proposto va in questa direzione e chiede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge,

La questione era già stata valutata in Commissione dove, giustamente, era stato rimarcato il fatto che il principio poteva essere condivisibile ma vi era il rischio che, nell'articolazione nelle diverse situazioni territoriali, si determinassero delle differenziazioni troppo rilevanti, che ci fosse il pericolo di una non sufficiente omogeneità. Siccome condivido questa osservazione ho riformulato l'emendamento, ribadendo l'obiettivo della definizione di un codice deontologico

in funzione dell'omogeneizzazione, definiti dall'Unione delle camere di commercio a livello nazionale, sentite le rappresentanze nazionali più significative degli amministratori di condominio. Mi auguro che questo emendamento, in coerenza con le cose che sono state proposte, venga diversamente considerato nel parere del relatore e del rappresentante del Governo. Grazie

alla normativa che viene innovata con questo provvedimento relativamente all'attività dell'amministratore di condominio, alle garanzie che i condomini devono assumere

Uno degli aspetti più delicati di questa riforma riguarda proprio la ridefinizione dei poteri, dei profili di responsabilità, del rapporto tra l'amministratore, i condomini e l'assemblea di tenuta della contabilità in modo corretto e tempestivo, la prestazione di garanzie che si è introdotta opportunamente con la prestazione di un'adeguata polizza fideiussoria. il principio della definizione di un codice di comportamento, deontologico, nei termini recati dall'emendamento

l'emendamento 26.101 tende ad introdurre un requisito per l'iscrizione nel registro degli amministratori di condominio

di scuola media superiore. Noi tutti sappiamo, per la ragione cui accennavo poco fa, quanto sia importante l'esercizio di questa funzione per poter garantire un ordinato e corretto svolgimento della vita dei milioni di condomini nel nostro Paese. introdurre un minimo di requisito di scolarità, che non è - attenzione - né la previsione di un albo, né la previsione di un esame di abilitazione e neanche un irrigidimento dei requisiti di accesso all'esercizio di questa attività, ma è appunto la previsione di un minimo di scolarità, quella che oggi è mediamente acquisibile

assicurare l'esercizio efficace di questa attività di rappresentanza e di cura di interessi, a volte consistenti (pensiamo ai supercondomini, ai condomini orizzontali, pensiamo agli amministratori di condominio che esercitano questa funzione per decine, se non centinaia di condomini)

vi sia la capacità di leggere, di analizzare, di interloquire, di rapportarsi alle norme, a volte complesse, contenute nella disciplina del condominio che stiamo riformando, del regolamento dei condomini, delle situazioni, a volte complesse sotto il profilo economico, dei rapporti giuridici che si pongono. Quindi, prevedere questa soglia minimissima di accesso all'esercizio dell'attività di amministratore di condominio mi sembra assolutamente ragionevole. Pertanto, chiedo al relatore e alla

Il relatore non può che convenire in linea di principio con la ragionevolezza di quanto sostenuto dal collega, irrisolvibile problema di fondo in termini dei potenziali rischi che il provvedimento andrebbe a correre. Infatti, nel momento stesso in cui andassimo ad ad introdurre, da ora in poi - perché vi sarebbe una sorta di sanatoria per il passato, nei limiti di chi da almeno da due anni svolge questa il requisito di un titolo di studio, che oltretutto è superiore a quello della scuola dell'obbligo, determineremmo comunque, nell'ambito di una professione non regolamentata, l'individuazione di un parametro specifico di riferimento particolarmente selettivo. Questo - ripeto, ripeto, al di là dell'assoluta ragionevolezza delle osservazioni del collega Legnini - potrebbe far qualificare quello che è il registro, ma albo non potrà mai diventare, alla stregua di albo. Questa è l'unica ragione per la quale il relatore

sulla preclusione che vi sarebbe all'introduzione di questo accesso. In realtà, in questo caso, non si introduce alcuna regolamentazione

a dare la possibilità ad ogni singolo condomino di procedere all'installazione di quelle che sono comunemente intese come fonti rinnovabili, o comunque delle infrastrutture per le stesse, senza dover

pertanto l'obiezione della 5a Commissione, che era preoccupata che fossero costretti a farlo anche

abbiamo intrattenuto una discussione sull'emendamento - che necessariamente va inserita nella riforma del codice civile in tema di condomini, perché

della copertura, perché è stata eliminata la questione, che oggi è stata oggetto di discussione in Commissione, relativa alle possibili ricadute onerose per gli appartamenti di proprietà degli enti pubblici. In questo modo, tale obiezione mi sembra superata, anche per la cancellazione dei commi 4 e 6, che erano stati oggetto

potrebbe essere superflua la disciplina che si vuole introdurre, perché già oggi il condomino ha facoltà di intervenire direttamente (si pensi, ad esempio, all'installazione di un'antenna televisiva) con dei limiti ben precisi;

il relatore e il Governo hanno sottovalutato - mi permetto di dirlo - la portata positiva di una norma di questo tipo. Dire che la norma proposta, di notevole semplificazione, prevedendo l'introduzione di una sorta di silenzio-assenso da parte dell'assemblea di condominio per l'installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti di produzione di energia alternativa, sostanzialmente non cambia nulla ed è pleonastica, mi sembra eccessivo. In realtà questa disposizione una norma davvero utile e positiva, che consentirebbe di accelerare e a volte di rendere concretamente possibile l'installazione e quindi la maggiore diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che si stanno diffondendo nei modi, nelle forme positive che tutti conosciamo.

all'installazione. Non capisco cosa si stravolge. Non capisco quali siano le ragioni che ostano all'introduzione di una norma positiva che produce altri effetti rispetto alla regolazione della vita

Grazie